La discussione sulla Convenzione di Istanbul ci mette però anche nella condizione di valutare come alle antiche forme di violenza - definiamole, in maniera terribile, tradizionali - se ne vadano aggiungendo e sommando delle nuove. Ed è sulle nuove che conviene aggiungere la nostra riflessione e le nostre considerazioni. Infatti, alle antiche, non ancora superate, si vanno aggiungendo forme di violazione figlie di consuetudini religiose antitetiche alle conquiste più elementari di libertà, tradizioni sociali che tengono la donna in diverse forme emarginata, usi tribali che vengono importati da alcune etnie di migranti: dall'infibulazione (casi tristi e drammatici a ripetersi che continuano anche nella nostra Italia) ai doveri matrimoniali imposti dalla famiglia. la Convenzione di Istanbul, che stiamo discutendo e che andiamo a ratificare, prenda in considerazione, tra le forme di violenza, quello che di nuovo appare all'interno dell'Unione e gli strumenti necessari per affrontare queste nuove forme di violazione, sottoscrivendo un principio che a mio parere è un valore in sé: il godimento delle libertà e dei diritti costituzionali in qualsiasi Paese dell'Unione non prevede violazioni nel nome della tradizione, di usi o di costumi e nemmeno nel nome di Tutelare le diversità culturali e religiose vuol dire innanzi tutto non consentire a chicchessia di calpestare i diritti dell'individuo e quindi della persona.

accanto alla Convenzione, dovremmo lavorare perché il Governo italiano e il suo Presidente del Consiglio difendano nel cuore dell'Unione europea, e dunque a Bruxelles, una sorta di tavolato di diritti comuni, che debba essere considerato un requisito fondamentale per tutti quei Paesi che intendano aderire all'Unione. Esistono già valori che devono essere condivisi quando un Paese fa domanda di accesso, rischiano di essere, in questo tempo, troppo generici e vaghi. Si tratta di quel tavolato che richiamava ormai alcuni anni fa (10 anni fa) Ralph Dahrendorf, quando chiedeva all'Unione europea di impegnarsi concretamente perché in un tavolato di diritti comuni ciascun Paese Paese godesse della possibilità di avere diritti di base condivisi. L'Europa non può ancora ritenersi soddisfatta da questo punto di vista. La seconda considerazione è stata già richiamata ieri da alcune colleghe senatrici, che sono intervenute prima di me: aumentare i fondi a disposizione dei servizi sanitari regionali

quanti subiscono violenze domestiche. Vi sono già alcune esperienze regionali che vanno in questa direzione, ma interessano alcune Regioni-tipo: sono esperienze che hanno funzionato e, se hanno funzionato,

ci consentirebbe di chiudere un cerchio di essere portatori in Europa di una misura di civiltà e di libertà che legherebbe la ratifica e l'adozione della Convenzione anche ad una serie di provvedimenti specifici.

onorevoli colleghi, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è stata approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati, e altrettanto sono sicura si accingerà a fare questo ramo del Parlamento. Ci fa piacere che tutto l'arco politico si sia unito nel desiderio di dare un segnale chiaro e forte su questo tema, ma non vorremmo che con tale ratifica qualcuno pensasse di avere già esaurito l'impegno sul tema dove, anche nel nostro Paese, invece vi è ancora tanto da fare. Anzi, sotto certi aspetti, l'impegno è appena iniziato. Ricordo che gli obiettivi della Convenzione, per citare testualmente i primi articoli sono: perseguire perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne; promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne. Si tratta di obiettivi importanti che necessitano di interventi non solo in un'ottica di previsione di ipotesi di reato, ma anche su temi non certo facili ed immediati, perché incidono su campi complessi che hanno a che fare non solo con la legge, ma anche e soprattutto con la cultura, la psicologia e con forme relazionali articolate e complesse. In questi anni il nostro Paese si è già dotato di importanti strumenti che vanno nella direzione della tutela dalla violenza di genere, ma altri saranno necessari al fine di intervenire su problematiche sociali e culturali. Non sarà facile, ne siamo coscienti, e purtroppo le cronache ce lo confermano quotidianamente. Cerchiamo pertanto di focalizzare l'attenzione e di indirizzare gli sforzi oltre l'odierna ratifica della Convenzione, che, per quanto nobile, resta un atto programmatico se non si agisce su piani fattivi. Nonostante il riconoscimento di fondamentali diritti civili, sociali e culturali a favore delle donne, la violenza fisica, psicologica e sessuale è ancora oggi una delle forme di violazione dei diritti umani più grave e più diffusa. Numerosi sono gli episodi di violenza commessi nei confronti di donne molestate, minacciate, violentate, stuprate, uccise, vittime di ogni tipo di violenza per il loro rifiuto a sottoporsi - lo sottolineo - ad irragionevoli dettami fanatico-religiosi, a matrimoni forzati, alle mutilazioni genitali, alla tratta di esseri umani. Ciò avviene anche nel nostro Paese. Ricordo che la violenza sulle donne non è un fenomeno tipico degli ambienti degradati e nemmeno tipica solo dei nostri giorni,

con la quale la Cassazione ha deciso che non è obbligatoria la custodia cautelare in carcere per coloro che, anche in gruppo, hanno stuprato o picchiato una donna,

Queste sentenze colpiscono anche l'opinione pubblica, che ritiene invece assolutamente odiosi simili crimini. Nell'ambito della valutazione dei contesti in cui nascono molte violenze e discriminazioni non può essere taciuto, al di là di considerazioni retoriche e buoniste, ma anzi deve essere onestamente riconosciuto che l'aumento esponenziale del fenomeno dell'immigrazione da Paesi con radici culturali diverse da quelle nostre tradizionali ha messo a dura prova le politiche di integrazione e, nel contempo, ha evidenziato l'improcrastinabilità di interventi sul piano giuridico e culturale volti a garantire il rispetto della legalità e dei principi del nostro vivere civile da parte dì tutte le comunità, anche con radici culturali diverse, L'inclusione delle comunità straniere nel nostro Paese, a qualunque etnia, religione e cultura appartengano, passa inevitabilmente attraverso la forza delle donne di aprirsi al confronto.

vi è un invito rivolto agli Stati a vigilare - lo sottolineo - affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto onore non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare alcun atto di violenza. C'è un punto della Convenzione che vorremmo però non fosse utilizzato per agire a livello sublegislativo, usando magari i presupposti della Convenzione per creare disparità al contrario. La Convenzione, infatti, impone linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere anche in materia di concessione dello *status* di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale. Non vorremmo che questo generasse, al contrario, una disparità, con prassi facilitatorie nelle quali la condizione femminile potrebbe essere ulteriormente sfruttata per ottenere benefici, senza giovare alla parità di genere, né alla promozione della condizione della donna.

passa anche dalla valorizzazione del suo ruolo e della sua figura, non solo come vittima, ma nel riconoscimento del suo valore all'interno della nostra comunità. Oggi, più che nel passato, le donne sono chiamate ad affrontare nuove sfide e la loro presenza sociale è indispensabile per contribuire a far esplodere le contraddizioni di una società organizzata quasi esclusivamente su criteri di produttività. Uno dei principi cardine che da sempre ispira la linea politica e programmatica della Lega Nord è, infatti, la protezione, valorizzazione e sviluppo dei nuclei familiari come istituzione base irrinunciabile per garantire la salvaguardia dei valori necessari per l'educazione dei figli. Non dobbiamo rinnegare la forza generata dalla nostra identità e dai valori di eguaglianza che nascono da tutta la nostra tradizione storica, con la consapevolezza che dignità e diritti sono elementi su cui non è possibile scendere a patti. Sarebbe ancora più vergognoso farlo sotto la maschera buonista del rispetto di quelle che vengono ipocritamente definite tradizioni, senza avere il coraggio di ammettere che si tratta invece di pratiche barbare, violente ed incivili.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, gentile Vice Ministro, credo anch'io che la seduta di oggi, come quella di ieri, sia un atto solenne del Senato della Repubblica con alto valore simbolico. Ciò mi induce - non me ne vogliate - ad iniziare con un brevissimo riferimento storico

che le Danaidi subiscono poi il matrimonio e uccidono, diventando a loro volta assassine dei mariti; Questo però è un altro capitolo. È una prima, modernissima rappresentazione, quella di Eschilo, della complessità delle relazioni di genere e dell'eterno conflitto fra valori universali e convenzioni politiche contingenti. Vedo il vice ministro Dassù e ricordo una bella giornata alla Farnesina, in cui si parlava di donne che osano, che devono osare, come ci disse Hillary Clinton in un messaggio videoregistrato.

di cui il femminicidio è l'atto estremo, è ormai un fenomeno universale, ha carattere diffuso e generalizzato e colpisce sia i Paesi avanzati che quelli

La comunità internazionale ha mostrato una sensibilità crescente verso questo tema. Chi parla verso la fine di questi ampi dibattiti ha l'obbligo della sintesi ed è esentato dal citare tutti i riferimenti legislativi. Istanbul, la stringente dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, che forse è il primo documento istituzionale ed internazionale in cui la violenza contro le donne viene riconosciuta come violazione dei diritti e delle libertà fondamentali.

giuridico omogeneo e completo, che possa consentire la protezione, la prevenzione e l'eliminazione di questo drammatico fenomeno. Io penso, colleghi, che violenza e libertà non possano stare insieme in nessun posto del mondo: a maggior ragione nei Paesi dell'Unione europea, a maggior ragione in un Paese come l'Italia,

Definirei questa situazione un caso di strabismo fra l'iniziativa politica - nazionale ed internazionale - e la società, che sembra non rispondere alle istanze di progresso e che ci impone, dunque, di agire e di capire meglio, cominciando dalle cause del fenomeno e dalle sue radici nel contesto nazionale. Abbiamo constatato che non c'è stato un miglioramento delle condizioni di vita delle donne, delle ragazze e delle bambine, che sono ovviamente la categoria meno protetta di fronte alla violenza di ogni tipo. Ciò significa che non si tratta solo di un problema legislativo, ma soprattutto - è stato detto da molti - di un problema culturale. Il testo della Convenzione esplicita questo tratto e ne declina i conseguenti impegni governativi, sui quali vorrei soffermarmi rapidamente. Nel preambolo si riconosce «la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere»

agli articoli 12, 13, 14 e 15 del Capitolo III - obbliga a promuovere questo cambiamento socio-culturale, fondamentale per progredire e necessario per superare la discriminazione, creando condizioni di reale parità. Sappiamo bene in quali luoghi e con quali strumenti è possibile fare tutto questo. I luoghi sono la scuola e l'università ovviamente, ovviamente, sedi elettive di produzione di un pensiero critico e indipendente. I luoghi però - lasciatemi dire - sono anche le televisioni, che in altre epoche della storia del nostro Paese hanno avuto anche il merito di collegare sul piano linguistico e culturale un Paese «troppo lungo», come dicevano gli arabi, e molto frammentato, mentre oggi rischiano di frenare lo sviluppo culturale della società italiana, riproducendo stereotipi di genere arcaici ed aggressivi, in maniera seriale. I luoghi sono anche i nuovi mondi della tecnologia avanzata, a cui hanno accesso costante principalmente giovani uomini e giovani donne, molti dei quali minori. In essi, soprattutto, va ricercato il difficile equilibrio fra la libertà di espressione individuale e la tutela dell'individuo stesso dalle numerose forme di violenza sociale e verbale. Infine, lasciatemi fare un ultimo riferimento alla famiglia, implicitamente evocata nel titolo della Convenzione di Istanbul come una forma subdola ed inattesa di violenza contro le donne - quella domestica, appunto - e che vorremmo e dovremmo restituire alla propria funzione educativa ed e, per certi aspetti, insostituibile, quale sede di produzione di modelli positivi. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, gentile Vice Ministro, la nostra responsabilità, dunque, oggi va ben oltre il valore simbolico dell'atto di ratifica è un primo passo per sostituire la retorica di genere con una solida cultura dei diritti, dei valori dell'uguaglianza e del rispetto della dignità della persona umana.

Nella nostra idea di Europa - credo che possiamo concordare su questo principio generale - violenza e libertà non possono in alcun modo coesistere, né per gli uomini né per le donne.

Nella qualità di uomini e soprattutto - lasciatemelo dire - di meridionali non possiamo non sostenere questi concetti e postulati che rappresentano la quint' essenza della nostra concezione tradizionalista della famiglia e della nostra visione ideale della donna, sia essa madre, moglie, sorella o compagna di lavoro o di vita. Le donne - non va dimenticato - rappresentano da sempre l'unità e la forza indissolubile delle famiglie. Nel nostro Paese solo con l'approvazione della legge n. 66 del 1996 la violenza carnale, gli atti di libidine violenti e gli atti osceni vennero riconosciuti come delitti contro la persona. purtroppo sono passati 17 anni e in Italia la maggior parte delle violenze sulle donne rimane ancora sommersa. Esiste, infatti, un divario tra le denunce per violenza sessuale e le donne che avrebbero subìto uno stupro. Questo perché le donne tendono a denunciare più facilmente i reati se subiti da estranei piuttosto che da persone conosciute. La donna, infatti, tendenzialmente vuole tenere unita la famiglia, costi quel che costi. Il fenomeno attraversa trasversalmente tutte le classi sociali, senza distinzione di età, razza o etnia ed è - l'avete ripetuto tutti - una delle maggiori cause di morte o di invalidità permanente nelle donne fino ai 50 anni. Basta ricordare che dal 2005 al 2012 ci sono state circa 900 vittime. È diventato È diventato un fenomeno quasi quotidiano, tant'è che sembra che passi come un fenomeno fisiologico. Ma così non è e non può essere. È ancora impressa

La violenza contro le donne è una piaga sociale che purtroppo ha sempre trovato nel nostro Paese terreno fertile, una piaga che non si può risolvere con la sola repressione: non ci sarebbero né risorse né personale a sufficienza. È indispensabile, quindi, un'educazione al rispetto della donna, che deve essere trasmessa in famiglia, a scuola e attraverso i *media*. È indispensabile modificare stereotipi e rappresentazioni della donna veicolati dai mezzi di comunicazione e dalle pubblicità introducendo codici di autoregolamentazione e linee di comportamento per garantire innanzitutto il rispetto della figura femminile. Bisogna che i procedimenti penali a carico dei colpevoli abbiano un'attenzione particolare da parte della magistratura, sia per evitare che la loro lunghezza contribuisca a mantenere aperte per troppo tempo ferite dolorose e, soprattutto, per evitare una attività di *stalking*, anch'essa ora sanzionata penalmente e che questa si possa tradurre in qualcosa di ben più grave. Per questo chiediamo che sia opportunamente sostenute le forze dell'ordine, che spesso rappresentano il primo baluardo di salvezza per le vittime. Si tratta di operatori altamente qualificati che devono conciliare tecniche investigative e norme procedurali con dei risvolti umani psicologici. Chiediamo che il tema della violenza contro le donne sia all'ordine del giorno di tutti i livelli istituzionali, soprattutto quelli periferici, municipali e di quartiere perché è lì che si consuma la violenza ed è là che le donne devono essere sostenute per denunciare i soprusi. Occorre potenziare la rete antiviolenza incoraggiando le vittime a denunciare e occorre disporre di personale esperto che possa dare un sostegno e un aiuto immediato alla donna che ha subìto un sopruso. La violenza sulle donne è ancora oggi fra le forme di violazione dei diritti umani una delle più gravi e diffuse nel mondo occidentale: i più recenti riconoscimenti in tema di diritti civili, sociali e culturali a favore delle donne non hanno tuttavia fermato, o quanto meno delimitato, il fenomeno della violenza fisica, psicologica e sessuale nei confronti del genere femminile. Sui temi etici e sulla famiglia l'Europa individua principi di riferimento, lasciando ai singoli Stati l'onere di declinare questi temi nella ratifica e nella legislazione ordinaria, nel rispetto della storia, della cultura e dei propri principi costituzionali. Questo nuovo trattato è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro legislativo completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. In conclusione, auspichiamo che la ratifica della Convenzione di Istanbul possa avvenire in forma unitaria e condivisa, anche per dare un segnale forte al nostro Paese di una volontà ferma e determinata di contrasto alla violenza contro le donne.

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante finalizzato a creare un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. Sin dalle sue prime pagine, nel preambolo, emerge lo spirito della Convenzione, là dove si riconosce che «la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi,

Un approccio che parta da quella dimensione sociale e culturale che per anni, anche in epoca contemporanea, è stata ritenuta quasi inevitabile, storicamente determinata, è ora invece indicato apertamente come responsabile di una realtà distorta. Non esiste relativismo culturale né indulgenza quando si parla di abusi. Dare un nome alle cose è il primo passo per identificarle e denunciarle. In questa prospettiva la Convenzione di Istanbul lo fa sin dall'inizio, dall'articolo 3, passando in rassegna le principali formule utilizzate per indicare generalmente violazioni, soprusi, maltrattamenti

o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». La vera novità è quella di rappresentare questo tipo di violenza come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. È prevista inoltre una serie di misure per il sostegno anche economico delle vittime di violenze, a partire dalla realizzazione dei rifugi fino all'esistenza di fondi per il risarcimento, e una politica di educazione, sensibilizzazione e prevenzione. Peccato, però, il testo approvato dalla Camera dei deputati non contempli alcuno stanziamento senza il quale sarà difficile dare seguito ai principi siglati. Resta inoltre il problema sostanziale dell'effettiva entrata in vigore della Convenzione, che avverrà avverrà il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione. Sarà quindi uno strumento monco se i 29 Stati firmatari non accelereranno le pratiche di ratifica che, ad oggi, riguardano solo Albania Montenegro, Portogallo e Turchia, sebbene la violenza sulle donne sia un fenomeno che investe tutta l'Europa, da Nord a Sud, da Est a Ovest.

Questi dati sono allarmanti e sono solo quelli emersi, essendocene molti altri nascosti dietro la paura. La Convenzione in esame, se attuata da tutti i Paesi membri, potrebbe salvare e cambiare la vita di milioni di persone e dare un contributo concreto al miglioramento del rispetto dei diritti umani e dello *status* delle donne. Per questo ne auspichiamo una celere e costruttiva approvazione, in quanto rappresenta una battaglia di civiltà a cui la politica e le istituzioni non possono e non debbono sottrarsi. Ma ciò non basta. Oggi, colleghi, qui e all'interno delle istituzioni, siamo chiamati ad affrontare una questione morale. Non si può infatti tacere di fronte alla violenza. Non possiamo denunciarla soltanto dopo che essa abbia avuto luogo. Non bisogna parlare solo di punizione del reato, solo del fatto compiuto. Dovremo riuscire ad attuare un vero cambiamento di rotta, attuando forme di prevenzione ed educazione ad una reale parità di genere sin dalle scuole, educando anche sul come denunciare e sul come proteggersi dalla violenza. L'obiettivo a cui guardare per generare un reale cambiamento sarebbe, infatti, promuovere nella società una reale acquisizione di consapevolezza della complessità e della dignità della persona in tutti i suoi generi. L'ostacolo da superare è la tendenza a ridurre ad oggetto di possesso, reale o virtuale, la bellezza dei corpi, soprattutto delle donne, sulla televisione, sul *web* e sui giornali. Tra tutte le persone rappresentate in pubblicità come oggetto, più o meno espresso, di desiderio e possesso, le donne sono forse quelle che pagano un prezzo maggiore. È appena il caso di rilevare che la pubblicità, per l'affinamento delle metodiche di persuasione e per la pervasività tramite giornali e televisione, costituisce oggi un elemento generatore di costume, forse il più forte. Ad essa si affianca la televisione commerciale, che degli stessi schemi si nutre e gli stessi schemi propone: corpi seminudi; ammiccamenti criptosessuali in cui il cibo e la donna vengono assimilati e le auto potenti sono viste come nasse in cui far impigliare giovani donne rappresentate come prede più o meno facili. In questo contesto antropo-culturale si genera non solo la rappresentazione e l'autorappresentazione delle donne come preda del maschio ricco o potente, ma anche la compressione della realizzazione del genere femminile. Se una donna vuole far carriera, dovrebbe o lasciarsi corteggiare dal maschio potente o competere con i maschi a spese della propria femminilità, con il sacrificio della maternità o della cura dei figli, atteggiandosi socialmente a maschio. Alla fine la singola donna riesce a vincere, ma la femminilità viene repressa e negata nei suoi aspetti che non si confanno al sistema produttivo. Tali variazioni del femminile nella cultura occidentale contemporanea sono andate ad innestarsi nelle rappresentazioni tradizionali della donna, ridotta a solo moglie o solo madre, predestinata quindi a sacrificarsi al successo anche a livello di immagine del nucleo familiare: concetti che sarebbero superati da decenni se non fossero stati reiniettati nel tessuto culturale da massicce dosi di *serial* televisivi di provenienza americana o latino-americana, propinati nel recente passato dalle televisioni commerciali e scelti per il loro basso costo. Il problema che si cerca di evidenziare è che la modifica dell'ordinamento, indotta dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, pur necessaria per arginare i fenomeni di violenza sulle donne, non è sufficiente se non trova una corrispondenza in una convergente modifica del ruolo sociale della donna, da definirsi in ambito etico e culturale in senso antropologico. La pari dignità dei generi deve diventare di moda; deve essere diffuso un giudizio di grettezza nei confronti dell'androcentrismo. A chi assegnare il compito arduo di promuovere tale profonda modifica della cultura? Quali le agenzie potenzialmente più efficaci? Noi ne proporremmo due: la scuola pubblica e i *media* di massa, tramite il servizio pubblico. Probabilmente, nessuno dei due elementi da solo mostrerebbe efficacia adeguata ma, opportunamente sommati e combinati, sono elementi che recentemente stanno dando buona prova, per esempio nella lotta contro l'omofobia. Il veicolo migliore, oltre ai programmi che stimolano il senso critico, sono probabilmente i programmi di intrattenimento, le *fiction*, che sembrano costituire un elemento trainante nella diffusione delle opinioni. Definita quindi una strategia di questo genere, appare credibile che le nuove norme possano trovare effettività non solo nelle sanzioni ma, prima e di più, nella progressiva introiezione dei relativi fondamenti etici nei costumi dei cittadini. In conclusione, quindi, il Movimento 5 Stelle propone di cogliere l'occasione della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per adottare un'azione multilivello orientata ad un mutamento reale delle condizioni delle donne in Italia, che costituisca premessa sufficiente per la lotta ai delitti contro di esse, ma anche alla cultura sottesa a tali delitti. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà. Signor Presidente, colleghi, siamo a un appuntamento importante che la Camera ha ha già avuto modo di approvare, peraltro con un dibattito intenso e importante, e il Senato oggi conclude questo percorso significativo per la storia delle donne, non solo italiane, e della loro aspirazione alla parità e all'emancipazione vera. Il preambolo di questa Convenzione riconosce e individua la grande importanza del tema della violenza, quella contro le donne, come una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, ed aspira a creare un'Europa libera da questa violenza. Ha ragione il collega Nencini, che prima è intervenuto con tanta passione e con riflessioni molto importanti: abbiamo tanta cura e attenzione ai numeri dell'Europa e alle regole dell'Europa, ma ci dimentichiamo spesso dell'Europa dei princìpi e dei diritti di cittadinanza. La Carta di Nizza e il Trattato di Lisbona, che il collega Nencini ha citato, sono la più significativa manutenzione costituzionale dell'Europa, quella che ancora dobbiamo costruire, e c'è tanta modernità e attualità nelle analisi del tempo - quelle che prima ricordava Nencini di Dahrendorf e, io aggiungo, quelle di Jacques Delors - sull'Europa libera Delors - sull'Europa libera da questa violenza. Il ministro Cancellieri ha ragione quando afferma in modo molto semplice che la violenza sulle donne è inaccettabile in una società civile; un fenomeno che continua a crescere in Italia, spia di una cultura atavicamente contro il femminile. È proprio da qui che dobbiamo partire e ripartire, e lo ha sottolineato benissimo la presidente della RAI Anna Maria Tarantola, nell'individuare nello sforzo congiunto nei luoghi di lavoro, in famiglia e attraverso i mezzi di comunicazione forse la strada da intraprendere. Ormai da tempo ci si interroga infatti su quanto la rappresentazione della donna attraverso i *media* e la pubblicità sia determinante nel rafforzare l'idea che la donna sia diventata una merce e il suo corpo considerato soltanto a livello sessuale e, come tale, una proprietà. Il CENSIS, nell'ambito del progetto «Women and media in Europe», ha realizzato un'indagine sull'immagine della donna nella televisione italiana, e da questa analisi emerge che le donne, nella fascia preserale, ricorrono nella nostra televisione pubblica, caro presidente Zavoli, soprattutto nei ruoli di attrici per il 56,3 per cento, di cantanti per il 25 per cento e di modelle per il 20 L'immagine più frequente della donna, quindi, è quella della donna di spettacolo, mentre, nei programmi di informazione, la donna compare soprattutto all'interno di servizi di cronaca nera, per il 67,8 o in vicende drammatiche in cui è coinvolta come vittima di violenze o di prevaricazioni di ogni tipo. La ricerca ha riguardato l'analisi delle leggi, i codici di autoregolamentazione e le buone pratiche riguardanti gli stereotipi di genere, attraverso la rilevazione presso le *Authority* e le principali emittenti televisive europee, da cui emerge che la tematica del contrasto agli stereotipi di genere viene assunta come grande impegno democratico e civile ma poi resta sulla carta. In Senato sono state presentate iniziative legislative contro il fenomeno del femminicidio da parte di tutti i Gruppi. Pochi giorni fa ne abbiamo condivisa una con la senatrice Mussolini, che introduce un'aggravante ai delitti contro la persona nei casi di violenza contro le donne. Ma tutti i Gruppi parlamentari hanno rivolto una lettera al presidente Grasso, su iniziativa della vice presidente Fedeli, nella quale chiedono che sia istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta che delinei questo orrendo fenomeno. Il Governo Letta ha istituito una*task force* interministeriale contro la violenza verso le donne e la figura di consigliere per le politiche di contrasto alla violenza di genere e al femminicidio. Considero questo un atto importante, che va nella direzione che auspicava prima il collega Nencini nel suo intervento. Ricordo anche, però, per verità, che durante il Governo Berlusconi, nel gennaio 2011, è stato siglato quel protocollo d'intesa tra il Ministero delle pari opportunità e l'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria che forse è l'unico atto formale che ancora oggi abbiamo. Tale protocollo prevede che gli operatori di pubblicità e i loro utenti «adottino modelli di comunicazione commerciale che non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne; tutelino la dignità delle donne, rispettando il principio di pari opportunità e diffondendo valori positivi sulla figura femminile; siano attenti alla rappresentazione dei generi e rispettosi delle identità di donne e uomini», coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società; «evitino il ricorso a stereotipi di genere» e favoriscano e rafforzino ulteriormente «l'applicazione del divieto di utilizzare l'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio» o tale da incitare alla violenza sulle donne. Tutti principi importanti, che non sempre sono attesi nel modo giusto, perché noi continuiamo a vederci proporre immagini che sempre di più le donne e le ragazze di oggi considerano stridenti con la loro cultura e con la loro evoluzione. Ecco perché occorre iniziare immediatamente un lavoro serio, per richiamare tutti al rispetto e all'applicazione delle norme che già esistono. Abbiamo l'obbligo di dare risposte vere ed efficaci ai cittadini, per non assistere più a episodi efferati come quelli riportati dalle cronache giornalistiche. Perdere altro tempo su questo fronte è davvero pericoloso per la democrazia e le sue istituzioni. I dati resi noti dall'ISTAT nel 2012, citati da molte colleghe intervenute prima di me, ci parlano ormai di una mattanza, non più di un fenomeno dai contorni fisiologici. Infatti, sono quasi 7 milioni le donne italiane tra i 16 i e 70 anni che hanno subìto nel corso della vita, dentro o fuori dalla famiglia, una forma di violenza fisica o sessuale; e 400.000 donne hanno subìto forme di violenza sessuale prima dei 16 anni; oltre 7 milioni di donne hanno subìto o subiscono violenza psicologica;

e in poco meno della metà di questi casi la violenza è perpetrata da un conoscente o da un parente. Le Regioni con le quote più elevate di donne che hanno subìto violenza fisica o sessuale da un uomo qualsiasi sono quelle del Nord e quelle del Centro, in particolare nei centri metropolitani (il 42 per cento). In Emilia-Romagna e nel Lazio le vittime sono oltre il 38 per cento della popolazione femminile; in Liguria il 35,4 per cento, a fronte di un valore medio nazionale pari al 31,9 7 per cento di coloro che subiscono violenze fisiche o sessuali dal *partner* le denuncia. Ciò è giustificato dal fatto che solamente una donna su tre le considera dei reati e forse questo è ancora l'aspetto più inquietante di questa vicenda. Le quote di donne che sporgono denuncia sono inferiori alla media nazionale non solo in tutte le Regioni del Sud, ad eccezione della Puglia, ma anche in alcune Regioni del Nord, come per esempio il Piemonte o l'Emilia-Romagna. Se ci si riferisce solo a stupri o tentativi di stupro, la percentuale delle donne che si considerano vittime di un reato sale al 26,5 per cento, ma le denunce restano limitate al 4,1 per cento nei casi di violenza. Concludo, Presidente, con una frase di Kofi Annan che a me sembra molto adeguata al voto di oggi: «I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano. Lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell'umanità. Il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l'umanità».

cara Vice Ministro, credo che la ratifica della Convenzione di Istanbul sia davvero un atto importante, che impegna questo Parlamento a realizzare misure concrete (come tutti hanno già in parte evidenziato, a partire dal finanziamento dei centri antiviolenza per i quali in seguito andranno assolutamente trovati i soldi)

I motivi per cui la Convenzione è il più avanzato strumento di contrasto alle violenze di genere sono stati ben presentati, secondo me, nell'ottima relazione della senatrice Fattorini e nella mozione unitaria che voteremo.

Gli stereotipi sono le immagini mentali con cui rappresentiamo la realtà. Sono semplificazioni rigide che usiamo come scorciatoie rispetto alla complessità del mondo. Sono costruzioni sociali che si radicano poco a poco, fino a diventare idee stabili che si tramandano tra generazioni, nelle famiglie, nelle scuole. L'uso degli stereotipi di genere produce una rappresentazione rigida, distorta e illiberale della realtà che si basa su ciò che ci aspettiamo dalle donne e dagli uomini. e dagli uomini. Sono aspettative consolidate che non vengono messe in discussione perché apparentemente fondate su differenze biologiche tra donne e uomini. Quelle aspettative, invece, sono rappresentazioni culturali che derivano dalle esperienze accumulate nel tempo. Gli stereotipi non hanno nulla di naturale, ma presentano il vantaggio di categorizzare, di rendere semplice ciò che è complesso. Sono una forzatura cognitiva, che elimina profondità, complessità e differenze. In Italia in particolare c'è forte resistenza nel superare un modello culturale maschilista che non concepisce le donne in posizioni di pari potere pur nel riconoscimento della differenza di genere. Anche nella famiglia, come dimostra la questione del cognome materno. E non è un caso se è proprio nei modelli di famiglia, in concezioni del rapporto di coppia fondati sulla gerarchia, in un'idea dell'amore come possesso che si nascondono, spesso subdolamente, non riconosciute, le ragioni culturali che portano alle violenze verso le donne, spesso - anzi, quasi sempre verso le donne amate. «Ti amo più della mia vita», viene detto; «Ti amo più della tua vita: e quindi o sei mia o ti uccido». Questo è falso amore. Le cose hanno iniziato a cambiare nella nostra società da quando il movimento femminista e femminile, vecchio e nuovo, ha proposto una diversa idea della donna, ha messo in agenda e nel dibattito la libertà, l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne. Ma adeguare il linguaggio e superare la banalizzazione delle scorciatoie cognitive è difficile e lento, e siamo molto, molto indietro. Il linguaggio è l'insieme dei modi con cui diamo senso alla realtà, la chiamiamo e comunichiamo. Nel linguaggio si formano e risiedono gli stereotipi. Nelle parole, nelle immagini, nelle emozioni che usiamo si annidano discriminazioni. Si annidano, si radicano, si tramandano. Perché nel terzo millennio è così difficile adeguare al genere il linguaggio? Si tratta di una questione di potere. Il mondo parla e si rappresenta visivamente al maschile, perché maschile è stata da sempre la storia della società. Faccio un solo esempio per farmi capire: se dico «il governante» ci viene in mente chi governa un Paese, ma se dico «la governante» viene in mente chi gestisce la casa. Il linguaggio, culturalmente radicato e cristallizzato in stereotipi, diventa così elemento di conservazione piuttosto che di progresso, di innovazione e di cambiamento. Una responsabilità notevole in questo senso ce l'ha il sistema mediatico e dell'informazione, che tranne poche eccezioni non ha saputo in questi anni fronteggiare il decadimento culturale e morale, che ha accentuato il peso degli stereotipi e delle discriminazioni di genere. Quando i mezzi di comunicazione riflettono il clima sessista nazionale senza contrastarlo, di fatto lo amplificano e lo legittimano. Ogni volta che ripropongono modelli femminili appiattiti, passivi e stereotipati, li consolidano. Vale per la televisione, per l'informazione, per la pubblicità. La pubblicità sessista non riguarda solo i corpi nudi. È quella che riduce le donne a pochi stereotipi ricorrenti e impoveriti. Non è sufficiente l'intervento del Gran Giurì. Bisogna lavorare preventivamente: servono regole, serve condivisione, serve un profondo e costante criterio di innovazione. Ecco perché voglio parlare anche di educazione, e concludo. L'intervento educativo è l'unico strumento che abbiamo per contrastare gli stereotipi restituendo alla nostra rappresentazione del mondo e dei generi profondità e complessità, uguaglianza e differenza. La scuola è l'unica possibilità che abbiamo per cambiare la mentalità e per costruire nuove donne e nuovi uomini; una società in cui la parola «femminicidio», a quel punto,

Però, come ho avuto modo di dire altre volte, diffido sempre di facili unanimismi e quindi vorrei sottolineare che

Lo dico perché questo non porta poi a risultati fattivi, concreti e confonde un po' le acque.

non sono tali ma significative di un approccio maturo, concreto, secco, reale e non buonista, come diceva il collega della Lega, che è ricorso spesso,

per vedere la prevenzione e la cultura, per puntare davvero sulla ricostruzione del tessuto delle relazioni in una società postmoderna che non ha la brutalità di un mondo islamico (penso

di risorse, poche ma certe, e di una struttura leggera, che non si aggiunga alla pletora di commissioni e organismi, ma che davvero abbia la funzione di drenare risorse e di intervenire con urgenza e nei tempi medio-lunghi.

un concreto, reale e fattivo *pressing* sulle sedi opportune, bilaterali e multilaterali, affinché gli altri Stati membri dell'Unione europea

vorrei dire poche parole a conclusione di una discussione che ho trovato veramente interessante e anche di grande livello. Penso non capiti tutti i giorni, né a voi né a noi quali esponenti del Governo, di ascoltare interventi così convincenti e di partecipare a un'azione collettiva così importante.

la relatrice, senatrice Elena Fattorini, e ieri le senatrici Bisinella e Mussolini, che hanno integrato la presentazione delle due mozioni. Queste ultime, a mio modo di vedere (nel merito ha già espresso il parere tecnico il sottosegretario Legnini), si completano; hanno accenti diversi, ma in realtà coprono i tre punti che a me sembrano fondamentali, cioè la prevenzione, la protezione e la punizione. Questi tre aspetti sono presenti, con accenti diversi sulle famose tre «P», in entrambe le mozioni. Ho ascoltato la replica della senatrice Fattorini e credo che come Ministero degli affari sia di mia competenza insistere su un punto: il nostro impegno affinché la Convenzione di Istanbul non rimanga sulla carta (un rischio che molti di voi hanno giustamente sottolineato), ma entri rapidamente in esecuzione.

sia in sede bilaterale che multilaterale, sui nostri *partner*. A quanto ci risulta - desidero comunicarlo a questa Assemblea - quattro Stati membri del Consiglio d'Europa si sono già impegnati a ratificare la Convenzione entro quest'anno:

potrebbe avere un effetto di trascinamento; in fondo, l'Italia è il primo grande Paese dell'Unione europea a ratificare la Convenzione è un tema chiave per i motivi interni che voi avete così bene descritto. Credo che la nascita di una *task force* sia un segnale importante della rapidità

Fattorini e da molti altri suoi colleghi, vi è un problema di fondi. Come noto, vi è un parere relativo alla neutralità finanziaria e dunque oggi votiamo la ratifica in regime di neutralità finanziaria,

la Dichiarazione di Vienna sul femminicidio: si tratta di una dichiarazione importante che verrà presentata come risoluzione alla prossima Assemblea delle Nazioni Unite. Infine, se posso unire i fili di questa discussione così interessante, credo di poter trarre due indicazioni generali, forse molto meno

questo è solo un punto di partenza. È un primo passo, come avete detto molto giustamente, che avrà davvero senso nella lotta alla violenza sulle donne se sapremo far seguire una serie di azioni concrete sia sul piano dell'adeguamento interno sia sul piano dell'iniziativa internazionale. Questo è un primo punto che mi sembra importante. che avete messo in luce molto giustamente è che l'azione contro la violenza sulle donne, sul piano interno ed internazionale, non può restare un'azione emergenziale - come è stato fino ad oggi

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, in sede di adozione dei provvedimenti esecutivi, vengano stanziate, ove necessario, le risorse finanziarie adeguate a garantire il puntuale rispetto degli impegni contenuti nella Convenzione».

che si è svolto oggi in Aula e anch'io considero la ratifica della Convenzione soltanto come il primo passo di un lavoro, soprattutto culturale, che dovremo fare per cambiare le relazioni tra generi.

società, proprio perché è determinata da fattori sociali, culturali ed economici, ed è una delle peggiori forme di discriminazione. È il modo con il quale gli uomini - come è stato detto - esercitano potere e controllo sulle *partner*: molti uomini credono, infatti, di avere il diritto di usare violenza fisica, verbale, emotiva e sessuale. Se dunque non ci sarà una condanna sociale netta, questi comportamenti continueranno ad esistere. C'è quindi una dimensione sociale della violenza, proprio perché essa riguarda tutti non soltanto le singole donne, ma le famiglie e la collettività intera, in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, senza tralasciare gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per tutta la società. La conquista dell'uguaglianza - è stato detto - ed il rispetto della dignità umana e della libertà della persona devono essere, quindi, obiettivi primari per l'intera società. Il testo della Convenzione su questo è molto chiaro, parlando proprio di prevenzione e contrasto. Noi pensiamo ad un insieme di interventi mirati, con un lungo lavoro sociale di prevenzione, formazione ed educazione. Confessiamo di non essere stati particolarmente attratti dall'ipotesi

non possiamo poi tralasciare la formazione per le forze dell'ordine, che spesso sono le prime ad essere coinvolte, anche se non sempre sono in grado di intervenire e percepire fino in fondo le dinamiche di contesti familiari complessi.

di libertà delle donne. Allo stesso modo, consideriamo interessanti le esperienze avviate in alcuni territori del nostro Paese di centri di ascolto per uomini maltrattanti, uomini che stanno riflettendo sui propri comportamenti, sulla rabbia, su problematiche relazionali, sulla genitorialità

proprio per un lavoro serio e concreto, in modo da riuscire ad incidere profondamente sul cambiamento, nell'assunzione delle responsabilità familiari uomo-donna e nel raggiungimento di una democrazia paritaria all'interno dei rapporti familiari ed affettivi. Non meno importante, come è stato ricordato, è il ruolo dei mezzi di comunicazione, che dovrebbero usare un linguaggio più rispettoso della dignità umana e delle figure femminili. Troppo spesso sentiamo, infatti, messaggi pubblicitari sbagliati nei palinsesti, nelle trasmissioni televisive nei titoli delle notizie, dove sessismo e omofobia prevalgono nell'esasperata esaltazione di quello che Lorella Zanardo ha definito molto bene ne «Il corpo delle donne». Si tratta di un impegno al quale, credo, nemmeno la politica possa più sottrarsi perché negli ultimi venti anni è stato dato un contributo negativo ai modelli culturali. Concludo dicendo che la Convenzione avrà un'importanza fondamentale e concreta per i meccanismi che saprà mettere in moto, perché vorremmo evitare che sia un'ennesima ottima enunciazione. Il paradosso che viviamo è che per due giorni in questa Aula abbiamo discusso

la firma e l'approvazione della Convenzione possa essere un segnale forte anche per aiutare la lotta di liberazione in atto in Turchia.

permette all'Italia di fare un ulteriore passo avanti nel contrasto alla violenza, contro ogni forma di violenza, ma con particolare attenzione a quella e nei confronti delle donne. tipo di violenza ha molteplici manifestazioni ed è una delle più vergognose tra quelle che ledono i diritti umani: cosa c'è di più brutale della violenza di un essere umano su un altro essere umano? Per questo continuerò a denominarla in tutto il mio intervento come «un crimine contro l'umanità» sul quale dobbiamo profondamente interrogarci. Già in vista della firma della Convenzione, il Parlamento italiano, nella XVI legislatura, aveva rivolto al Governo numerosi atti di indirizzo. Voglio ricordare brevemente che lo scorso 20 settembre 2012 il Senato aveva approvato un ordine del giorno e sette mozioni, che impegnavano il Governo a sottoscrivere la Convenzione di Istanbul e ad attuare quanto in essa previsto, anche in seguito alle risultanze del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne riguardanti il nostro Paese. Non voglio cimentarmi nel consueto elenco delle donne che in questi anni, mesi o giorni hanno subìto violenze o, a causa di queste, hanno addirittura perso la vita; sono tante, sempre troppe, ma relegarle ad un banale elenco non serve né a loro né alla nostra società. Credo invece utile rinnovare gli obiettivi da mettere in campo da parte delle istituzioni, delle associazioni, dei *media* e non meno del mondo della scuola e della cultura. importante promuovere un mutamento radicale di mentalità, attraverso l'affermazione di un pensiero nuovo che impedisca la riduzione della persona ad oggetto, così come richiede la Convenzione stessa; stessa; dobbiamo infatti ricordarci che il problema della violenza sulle donne non è un residuo del passato e non va sottovalutato. Accanto agli atti di aggressione fisica e psichica bisogna poi combattere tutti quei fenomeni che causano la continua erosione della dignità femminile. Sul tema del contrasto della violenza sulle donne l'Italia comunque non parte da zero. La legge n. 38 del 2009 ha introdotto nel nostro Paese il reato di *stalking*, che incorpora già buone prassi per combattere gli atti persecutori, come previsto dalla Convenzione che ci apprestiamo a ratificare. Evidenti però sono ancora le carenze dello Stato di fronte ad un calvario di minacce e di violenze: spesso le donne si trovano davanti alla lentezza della burocrazia del sistema giudiziario. In questo percorso ad ostacoli il caso si perde e la denuncia va in prescrizione, con il risultato che la vittima rimane sola. Per questo occorre partire dai dati, che possiamo reperire anche tramite le forze dell'ordine e le associazioni che operano sul fronte del contrasto alla violenza sulle donne,

Permettetemi, dunque, di dire che ho accolto favorevolmente l'impegno del Governo a trattare il fenomeno della violenza sulle donne agendo in sinergia tra i diversi Dicasteri con piani ed azioni ben precisi: la promozione di un tavolo interministeriale per la predisposizione di progetti coordinati per tutto il territorio nazionale, così da garantire una maggiore incisività nel contrasto alla violenza di genere, e non meno l'istituzione di un Osservatorio nazionale permanente sulla violenza alle donne» (di cui, voglio ricordarlo, si parla da anni), che sicuramente è un'iniziativa da prendere in seria considerazione. Confido quindi, nell'impegno dichiarato fin da subito dal presidente del Consiglio, Enrico Letta, dal ministro Alfano, dal ministro Cancellieri ed dal ministro Idem. Ministro, desidero rivolgere un particolare apprezzamento per l'importante risultato ottenuto con il recente incontro che ha promosso per ascoltare la base, o o meglio tutto quel mondo insostituibile formato dalle associazioni femminili e non meno dai volontari, dai rappresentanti delle scuole, del comparto sanitario e delle forze dell'ordine, quotidianamente impegnati in prima linea nel prevenire e combattere la violenza sulle donne e sui minori. Desidero a tal proposito comunicarle, signora Vice Ministro, che essendo già da tempo in contatto con i responsabili del settore sanitario che hanno attivato i presidi in Rosa nei Pronto soccorso, sto valutando con loro alcune azioni - che le proporrò

Infine, dichiarando il voto favorevole del Gruppo GAL, desidero sottolineare tre priorità che mi stanno particolarmente a cuore. La prima riguarda la promozione di un precisa campagna culturale attraverso i mezzi di comunicazione, ma non meno mediante percorsi formativi da attuare nelle scuole di primo e secondo grado che possano vedere coinvolte le forze dell'ordine competenti in materia per informare e sensibilizzare i nostri giovani. Su questo punto so che le ministre Idem e Carrozza si sono già espresse positivamente. la creazione di un giudice di famiglia che si possa occupare esclusivamente delle notizie di reato riguardanti la violenza di genere, i maltrattamenti in famiglia, le lesioni personali, l'inosservanza degli obblighi famigliari e di tutti gli atti persecutori. In sostanza, sarebbe un pubblico ministero istituito presso ciascuna procura, così da ottenere decisioni più rapide ed incisive in merito a misure di tutela della vittima e dei suoi famigliari. Anche sotto questo aspetto conosco la grande sensibilità del ministro Cancellieri e del ministro Alfano.

un fondo preciso e vincolato per il sostegno di centri antiviolenza e per promuovere, là dove occorra, il reinserimento della donna che ha subìto violenza, sostenendola quindi anche economicamente; senza soldi, signora Ministro, non si possono aiutare le donne a ricostruire il loro futuro e molto spesso a denunciare il proprio marito. Tutti questi passaggi la Convenzione di Istanbul li promuove; ora sta a noi, tutti insieme, attuarli concretamente. Signor Presidente, signora Ministra onorevoli senatrici e senatori, è difficile aggiungere qualcosa a tutto quanto è stato già detto in questi due giorni di autorevoli interventi che mi hanno preceduto e in cui in pratica sono stati toccati tutti punti

Come hanno dimostrato gli ultimi avvenimenti, sono ancora più gravi, assurdi e difficili da comprendere quando a compierli sono ragazzi giovani dico dovrebbero - avere assimilato le regole basilari del rispetto e della tolleranza, che dovrebbero essere insegnate dalle famiglie e soprattutto dalle istituzioni scolastiche.

all'informazione e all'educazione rivolta soprattutto ai giovani. Sono questi argomenti di importanza capitale per poter tentare di risolvere alla radice questo grave problema di distorsione, purtroppo, di tante culture e tanti popoli. Occorre entrare nelle scuole il più presto possibile, per incidere in modo efficace nella mente dei bambini contro modi di pensare e considerare le donne retaggio di mentalità arretrata e ormai superata, purtroppo

Ho avuto l'onore in Valle d'Aosta, in qualità di assessore, di presentare e far approvare in consiglio regionale la legge contro la violenza sulle donne, e altre Regioni in questo senso si sono mosse. Le ASL, da anni, hanno messo in piedi sistemi di accoglienza per le donne oggetto di violenza e i loro bambini. Non siamo quindi all'anno zero, ma sicuramente la ratifica di questa Convenzione rappresenta un ulteriore passo avanti verso il pieno riconoscimento e la piena tutela della donna della nostra società moderna. Signor Presidente, signora Ministro, signora Vice Ministro, onorevoli colleghi, oggi finalmente siamo alla ratifica di un'importantissima Convenzione, quella di Istanbul, volta a prevenire e contrastare i femminicidi, gli stupri e le altre forme di violenza di genere. Nel contrasto alla violenza sulle donne l'Italia - lo hanno ricordato anche altri colleghi che mi hanno preceduto - è tra i primi della classe, almeno sulla carta. Dopo che martedì 28 maggio la Camera ha approvato questa Convenzione all'unanimità, tocca a noi colleghi del Senato confermare questo impegno forte di volontà e di azione. Ringrazio anche i colleghi uomini che sono intervenuti nel dibattito e in fase di dichiarazione di voto per sottolineare come questo sia un drammatico problema che deve essere affrontato da noi tutti nella società. società. Le pagine di cronaca degli ultimi tempi riportano infatti con troppa frequenza - direi anzi pressoché quotidianamente - episodi di violenza contro le donne perpetrati nella maggior parte dei casi in un contesto familiare e domestico da parte di uomini che sono padri, fidanzati e mariti. Nell'anno passato sono state più di 120 vittime e ad oggi il loro numero è impressionante ed è ancora aumentato; questo è inaccettabile. Il fenomeno che oggi ha acquisito visibilità nei giornali in tutta la sua drammaticità, purtroppo non è occasionale o appena nato, ma finalmente viene ora analizzato nella sua specificità. La circostanza per cui i delitti sono commessi principalmente da un uomo che ha, o ha avuto, una relazione di affetto o conoscenza con la donna, la donna, esplicita una dimensione sociale della violenza, ancor più preoccupante per il fatto che le mura domestiche sono spesso la scena del crimine. Questo fenomeno si è rivelato di così grande portata da giustificare la scelta di coniare il termine specifico «femminicidio», per indicare la violenza misogina dell'uomo nei confronti delle donne «in quanto donne», introducendo un'ottica di genere nello studio dei crimini. È di fondamentale importanza provvedere in tempi rapidi alla ratifica di tale Convenzione, perché al momento - vorrei ricordarlo - essa non è ancora in vigore; noi saremo il quinto quinto Stato, dopo Albania, Portogallo, Montenegro e Turchia, ad averla ratificata (e in questi giorni parlare di Turchia che ratifica e propone una Convenzione come questa, con ciò che lì sta accadendo, fa pensare). Rimangono però ancora venti Stati, tra cui Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Svezia, che, pur avendo firmato il Trattato, non lo hanno ancora ratificato. Serviranno comunque le ratifiche di altri cinque Stati prima che la disciplina internazionale possa entrare in vigore, per questo è importante accelerare.

che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione», tale violenza ha natura strutturale, essendo basata sul genere ed «è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini». A livello poi di definizione, la violenza sulle donne viene ritenuta una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. La cosa importante è che il Trattato internazionale pone una serie di obblighi in capo agli Stati, affinché adottino politiche coordinate

costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini», in particolare sostenendo campagne di sensibilizzazione e - mi piace sottolinearlo - prevedendo anche programmi scolastici adeguati, incentivando l'informazione e i *mass media* ad elaborare norme di autoregolamentazione La Convenzione prende infatti in considerazione una serie di comportamenti violenti nei confronti delle donne e obbliga gli Stati a punirli, il più delle volte anche agendo a livello di ordinamento penale; vengono elencati lo *stalking*, la violenza fisica, lo stupro, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali, l'aborto o la sterilizzazione forzati, le molestie sessuali. Gli Stati devono prevedere il risarcimento delle vittime in ogni caso e la possibilità, in caso di matrimonio forzato, di invalidare l'unione senza oneri eccessivi per chi denuncia. delle disposizioni di carattere procedurale, basate soprattutto sull'individuazione di misure di protezione delle vittime: questo è un aspetto fondamentale, troppo spesso - e lo dicono le cronache quotidiane dei femminicidi - la violenza si sarebbe potuta evitare sterilizzandola sul nascere, se solo si fosse agito più velocemente. La Convenzione dispone poi che i reati in questione vengano perseguiti anche senza la denuncia da parte della vittima. Se una denuncia c'è, ma poi viene ritirata e le accuse ritrattate, lo Stato deve prevedere che il processo possa continuare. L'importanza di norme come questa si è vista anche di recente, ad esempio nel caso della giovane di Caserta, che ha prima denunciato e poi perdonato il suo persecutore. Al di là del volere della vittima (che spesso è vittima anche da un punto di vista psicologico), lo Stato, anche il nostro, deve poter proseguire il processo. Dunque, la Convenzione che ci accingiamo a ratificare si pone in buona sostanza l'obiettivo di proteggere le donne da ogni forma di violenza e di contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione, anche dal punto di vista giudiziario. Ma le parti del Trattato a mio avviso più importanti e sulle quali vorrei e sulle quali vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sono quelle - se ben recepite - di carattere più culturale, dove si chiede di intervenire nelle scuole, nei *mass media*, nell'educazione in generale, per fare quei passi avanti ancora necessari all'affermazione di un'immagine non discriminatoria della donna. Significativa, infatti, è l'ultima parte del trattato, dove si prevede che gli Stati eleggano, entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione, un organismo incaricato di vigilare sull'attuazione della stessa. Si tratta del

disponibili sono quelli ricavati dalle notizie riportate sui giornali, dato che non esiste un osservatorio preposto a monitorare questo fenomeno sommerso. Pertanto, con l'istituzione di questo organismo, l'Italia sarà costantemente monitorata nei suoi progressi nella lotta alla violenza contro le donne, e questo rappresenta un significativo passo E se sul piano della legislazione penale gli strumenti già esistono, sarebbe allora compito della politica concentrare i propri sforzi sull'affermazione di un diverso modello culturale. La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi e uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette spesso in una posizione subordinata rispetto agli uomini anche dal punto di vista economico. Dunque, l'elemento chiave per prevenire tale fenomeno, a mio avviso, è il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de iure*, ma anche *de facto*. Noi speriamo davvero che la ratifica di oggi sia un ulteriore passo verso questo obiettivo, che deve essere l'obiettivo principale, ossia far maturare la coscienza e la conoscenza la conoscenza del fenomeno drammatico che è presente nella nostra società, e che dunque possa contribuire ad accrescere la consapevolezza in tutte le istituzioni e nella società civile dell'effettiva natura del problema. Solo con un vero cambiamento, prima di tutto culturale, può essere sconfitto il terribile fenomeno del femminicidio

Varie sono le problematiche aperte che vanno affrontate. Il Governo, lo abbiamo sentito in questi giorni, da un lato afferma impegni importanti e condivisibili sul tema, poi però, andando nello specifico, si riscontrano alcune contraddizioni, ad esempio laddove è evidente che vi sia necessità di finanziamenti e contributi per chi sul territorio, a livello livello locale, si occupa della promozione delle pari opportunità e dei diritti di genere. Mi sembra, allora, una clamorosa contraddizione rispetto alle dichiarazioni di intenti: il Governo deve assumere come priorità il finanziamento di questi progetti e servizi contro le violenze di genere, altrimenti i discorsi che stiamo facendo su politiche e culture rimangono senza senso. È necessario, poi, oltre a prevenire, punire in maniera severa, applicando la pena in maniera rigorosa e dando applicazione ai principi dell'effettività, dell'efficacia e della certezza della pena. Altro che svuotacarceri, colleghi! È necessario che si applichino i provvedimenti restrittivi fin dal primo allarme, perché poi quasi sistematicamente si sfocia nella violenza. Occorre finanziare anche le reti di supporto, sostegno e divulgazione della cultura del rispetto della donna. In buona sostanza, questo rappresenta un passo avanti che aiuta a combattere quella che può davvero chiamarsi, a mio avviso, sottocultura del possesso, che toglie valore alla vita delle donne. Nel 2013, un Paese che conosce e vive quotidianamente la brutalità del dominio fisico, psicologico, di troppi uomini sulle donne, non può essere definito civile.

alla votazione del disegno di legge n. 720, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. Il nostro Paese ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012, con la dichiarazione esplicita che sarà applicata nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali e, nella fattispecie, dell'articolo 3, lettera *c)*, della Convenzione stessa. Lo strumento della Convenzione rappresenta il livello più avanzato dello *standard* internazionale di prevenzione e contrasto del complesso fenomeno della violenza sulle donne e di protezione delle vittime. In linea con la formula tipica dei trattati europei sul contrasto di speciali forme di violenza e abuso, il riferimento è ai tre momenti costitutivi dell'architettura garantistica convenzionale, e dunque alla prevenzione, alla protezione e sostegno delle vittime e alla punizione degli autori delle violazioni, corredati e rafforzati da una serie di altri impegni di carattere politico e sociale, finalizzati alla realizzazione di strategie integrate per il contrasto e l'eliminazione della violenza contro le donne e della violenza domestica. Tali reati, comunque, appaiono già in gran parte sanzionati dal codice penale nell'ambito dei delitti contro l'incolumità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, talvolta sotto un diverso *nomen juris*. Nell'ambito della comunità internazionale, l'ordinamento italiano si colloca tra quelli che già assicurano un elevato grado di conformità alla Convenzione, anche sotto il profilo della tutela penale. Ciò, evidentemente, non significa che nella nostra società la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica siano reati residuali. Cronache recenti hanno evidenziato la frequente drammaticità, la cui enumerazione statistica non si esaurisce nell'esigenza di una mera ratifica ed esecuzione della Convenzione in oggetto: sono ferite sociali. Non è forse inscritta nei diritti fondamentali di ogni essere umano la tutela della vita e della sua intrinseca dignità? Necessita ancora oggi affermare l'intollerabilità della violenza contro le donne? Si richiede una Convenzione che novelli, quanto già immediatamente e tangibilmente evidente, l'insopportabilità di tali crimini? Esistono, forse, crimini contro la persona più sopportabili ed altri meno? Ogni azione svolta con la forza, fisica o psicologica, finalizzata alla prevaricazione sull'altro, fino a togliere la vita, è sempre e comunque inaccettabile e insopportabile. Mi pongo altri interrogativi: la ratifica di una Convenzione può rappresentare una svolta concreta, almeno auspicabile, a una deriva sempre più evidente? Quante convenzioni, protocolli, carte europee, raccomandazioni, patti internazionali, statuti fanno da preambolo al testo della Convenzione di Istanbul, eppure i risultati ottenuti Riteniamo che, con la ratifica e l'esecuzione della Convenzione in oggetto, abbiamo pienamente soddisfatto il nostro ruolo di legislatori? La Convenzione - ultima e non secondaria domanda - può rappresentare lo snodo per una cultura sociale, pienamente avvertita e vissuta, che riconosca alla donna quanto riportato agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione? Prima di dare una risposta, ancorché parziale, ai predetti interrogativi, una premessa è necessaria al fine di fugare incerte interpretazioni: il disegno di legge, finalizzato alla ratifica della Convenzione, deve essere approvato.

ripetutamente afferma - dico giustamente - princìpi e valori che devono sostanziare il vivere dove non ci sia prevaricazione e sopraffazione, e non ci sia violenza ancor più nei confronti di coloro che - in un certo qual modo - si trovano in situazioni di particolare fragilità. Eppure, nonostante la pluralità di convenzioni, norme, leggi, dichiarazioni e trattati, le violenze contro le donne (e non solo) continuano ad essere cronaca dei nostri giorni: punte di *iceberg*, per la gran parte sommersi. Si richiede pertanto la comune consapevolezza che, pur avvalendosi del ruolo dissuasivo, punitivo e pedagogico della norma, necessita una concreta azione culturale volta al riconoscimento dell'intrinseca dignità femminile. Ritengo che l'azione della comunità non debba né possa limitarsi alla mera applicazione della Convenzione. Il dibattito odierno pone all'attenzione di noi tutti il devastante vuoto interiore che genera spregio della vita propria e altrui, supportato da un riduzionismo antropologico che dalla visione globale della persona vira alla sola dimensione corporea, biologica, meccanicistica, riduzionistica, in cui le scelte sono guidate dal semplice "sentire", vale a dire un assoluto da soddisfare. E in omaggio a questo *totem*, quante donne violate, quante vite distrutte, quante ferite aperte e dolenti, quante sconfitte irreparabili. Se la Convenzione sarà recepita - in condivisione politica, sociale e culturale - come espressione sostantiva della dignità femminile, come accoglienza e cura proprie del mondo femminile, si può sperare che favorisca lo sviluppo di percorsi educativo-formativi, nei quali la coniugazione complementare maschile-femminile rappresenti incontro e non possesso, e non dominio.

Signora Presidente, signore colleghe e colleghi, desidero iniziare il mio intervento esprimendo particolare soddisfazione per il fatto che il Parlamento italiano abbia inteso inserire tra i primi lavori di questa legislatura la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Istanbul, vale a dire il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che istituisce, nel quadro del Consiglio d'Europa, un meccanismo di tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, includendo la prevenzione, la repressione ma anche, aspetto non secondario, l'assistenza e la protezione delle vittime. Come ha avuto modo di precisare la relatrice in Commissione affari esteri, la senatrice Fattorini, a cui va il plauso per la puntuale e preziosa esplicazione, questo documento rappresenta il punto più avanzato del diritto internazionale sul tema, nonché il primo trattato che riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione, configurandola dunque come violazione del principio di uguaglianza tra i sessi. Finalmente si è chiusa un'era arcaica e brutale. Il mondo occidentale, traino giuridico mondiale da secoli, che sbandiera la sua superiorità nel riconoscere diritti civili e principi etico-morali di portata assoluta, ha deciso finalmente di dotarsi di strumenti giuridici adeguati volti a fronteggiare una moderna piaga sociale che sta caratterizzando tristemente gli inizi di questo millennio: la violenza in ogni sua forma nei confronti dei soggetti più esposti e maggiormente incapaci di difendersi e reagire. La *ratio*, la struttura legislativa, gli obiettivi e la necessità etica di questa norma sono stati individuati in maniera chiara e dettagliata. E questo è un grande segnale di civiltà, ma soprattutto è una presa di coscienza collettiva della comunità internazionale del fatto che questo fenomeno andava disciplinato nel più breve tempo possibile e nel più deciso e incisivo dei modi. Tra i principali aspetti vogliamo sottolineare una peculiarità di questa norma, di cui non è mai retorico parlare, soprattutto alla luce degli agghiaccianti fatti di cronaca quotidiana che vedono protagonisti e vittime donne e purtroppo bambini, perseguire non solo il fine di proteggere legislativamente le donne da ogni forma di violenza e contrastare la disumanità della violenza domestica, ma anche di contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le stesse e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione della donna in quanto tale. questo sia un aspetto della Convenzione molto importante su cui riflettere. Per troppo tempo si è affrontato il problema dell'assoluta e compiuta parità tra uomo e donna, anche in questo Paese, con molta superficialità, come è avvenuto per altre questioni sociali. Ci auguriamo che, recependo nel nostro ordinamento giuridico questo centrale complesso normativo internazionale in tema di protezione delle donne, l'intera concezione sociale in Italia sulla parità sostanziale uomo-donna trovi il suo fondamento valoriale e il suo faro legislativo. Spesso in passato - e non bisogna certo insegnarlo a noi italiani, figli del corpo giuridico del diritto romano - dal nucleo etico di norma giuridica la società ha tratto e sviluppato un senso comune e un codice comportamentale positivo ed innovatore. Il fatto che saremo il quinto Paese membro del Consiglio d'Europa a ratificare la Convenzione ci deve solo inorgoglire. I Paesi nordeuropei, in special modo nel mondo anglosassone, seguendo stereotipi storico-mediatici e di natura preconcettuale, guardano agli italiani ancora come ad un popolo legato ad antiquati ed anacronistici schemi familiari maschilisti nei quali emerge la figura del padre-marito padrone. Sappiamo che non è così, generazioni ormai, ma all'estero hanno una percezione diversa. Dare questo segnale, evidentemente di segno opposto, significa svincolarsi finalmente da questa immagine antica di famiglia mediterranea nella quale la donna riveste un ruolo solo marginale. Tuttavia, non possiamo negare che la violenza che affolla la cronaca nera dei *media* nazionali è figlia di una insufficienza culturale contro la quale è opportuno intervenire in maniera tempestiva. Le istituzioni di questo Paese hanno il dovere di impegnarsi fattivamente per creare le migliori condizioni giuridiche volte a combattere ogni forma di soppressione della volontà e della libertà individuale della donna. Noi parlamentari dobbiamo schierarci trasversalmente e senza esitazioni quindi contro tutti i profili di passività morale e materiale a cui vengono sottoposte le donne italiane e contro le "prigioni dell'indifferenza" entro le quali alcuni beceri individui relegano le proprie mogli, le ex mogli, le fidanzate, le ex fidanzate, le sorelle, le parenti, le amiche. passività che si manifesta nell'imposizione delle regole sociali della tradizione, nell'invadenza nelle scelte di vita fino alle forme più barbare di soppressione della volontà e conseguente violenza fisica e sessuale. Questa passività innaturale, l'incapacità di ribellarsi, l'assenza di condizioni e sostegni assistenziali per reagire ai soprusi poi produce la diffusa accettazione culturale della violenza. È lì che lo Stato, con gli strumenti legislativi e strutturali adeguati, deve intervenire, valorizzando le risorse, le competenze e le professionalità che ha a disposizione. attraverso le leggi, della fase della protezione sociale dei soggetti più esposti, diventa complice del carnefice materiale. Un importante strumento di innovazione legislativa in tal senso, in questi ultimi anni, si è rivelata la legge sullo *stalking*. Non è bastata. La cronaca ci dice che bisogna fare di più per difendere le donne La Convenzione servirà a questa innovazione culturale sostanziale. Tra i suoi obiettivi c'è da soffermarsi su quello della rivisitazione di tutto il sistema di prevenzione e di informazione scolastica prima, e mediatica poi, sul problema. È un ulteriore aspetto su cui puntare i riflettori normativi in seguito alla ratifica. Sul piano dell'educazione al rispetto della figura della donna si gioca una partita fondamentale. Molte aberrazioni che abbiamo letto sui giornali negli ultimi giorni, relative ai femminicidi più efferati, nascono dall'*humus* culturale della mancata considerazione della volontà di autodeterminazione della donna. In questo quadro delirante di valori, un diniego sessuale o sentimentale costituisce il presupposto per l'annientamento fisico di una persona, quasi non più considerata come tale, ma alla stregua di una cosa inanimata, priva di volontà individuale, indegna di riguardo collettivo e riconoscimento sociale. Con l'auspicio che il recepimento e l'attuazione di questo provvedimento possano costituire solo il primo passo o quanto meno la pietra miliare su cui innervare sostanza legislativa alla necessità storica della reale parità uomo-donna, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

signori senatori, signor Ministro, ci accingiamo a deliberare su un disegno di legge che riguarda finalmente le donne, su cui c'è il plauso convinto ed unanime del Gruppo del Popolo della Libertà. Lo sottolineo: le donne. Non è una banalità, non è una questione semantica, è una grande novità e lo voglio spiegare. Recentemente sono state approvate norme che possono essere considerate i precedenti di questo intervento di contrasto alla violenza alle donne, perché in Italia, come è stato qui sottolineato, non siamo all'«anno zero». Penso al decreto-legge n. 11 del 2009 contro la violenza sessuale e gli atti persecutori: ebbene, dei 14 ampi articoli di quel decreto-legge, l'unico che riguardi le donne è quello che aumenta la pena del colpevole di atti persecutori a danno di una donna in stato di gravidanza. Trattandosi di gravidanza, non si poteva non fare riferimento ad una donna! Per tutto il resto, gli interventi normativi riguardano la persona offesa, un'astratta persona offesa, che nella grandissima totalità dei casi è ovviamente una donna. Ricordo ancora, per esservi spesso intervenuta con il vigore e la convinzione che ho ritenuto necessari, il tema delle pari opportunità in materia elettorale. Ricordo - senza particolare piacere - il «pudore lessicale» che si è reso necessario, il riferimento a concetti neutrali come «nessuno dei due sessi» o a «candidati di sesso diverso», perché altrimenti si sarebbe violato - viene da dire paradossalmente - il principio Quindi, si interviene per riequilibrare una situazione clamorosamente sperequata a svantaggio delle donne, ma non si può utilizzare la parola donna o, se si usa come nella Costituzione, agli articoli 51 e 117 che abbiamo riformato, non si può scrivere da sola, ma nella formula «parità tra donne e uomini». Anche nel codice delle pari opportunità, queste sono - appunto - le «pari opportunità di uomini e donne». Insomma, quando si promuovono le pari opportunità, le donne sono sempre affiancate dagli uomini (cosa che posso anche capire), ma quando si tratta di violenza, le donne che la subiscono gli uomini li hanno di fronte. Sarà scontato, ovvio, evidente, ma è significativa la chiarezza con cui emerge nei testi al nostro esame che sono solitamente gli uomini ad uccidere e a percuotere le donne e non il contrario. Dati drammatici evidenziano che ogni giorno in Europa sette donne sono uccise dai loro *partner* e che nello scorso anno, in Italia, sono state uccise più di 120 donne, più di 120 donne, praticamente una ogni tre giorni: si tratta di una vera e propria mattanza! Ecco la semplice ma straordinaria novità di questo disegno di legge e della Convenzione che con esso viene ratificata: contiene settanta volte la parola donne e 70 volte la parola finalmente. Come ho già evidenziato, non è una questione semantica, ma un vero salto di qualità, che si misura già in quella parte del preambolo che, dopo aver riconosciuto la natura strutturale della violenza contro le donne come violenza di genere, riconosce anche che le donne sono esposte ad un più alto rischio di violenza di genere degli uomini. Di conseguenza, l'articolo 3 della Convenzione definisce la violenza di genere contro le donne come la violenza che è diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne sproporzionatamente. È un dato incontrovertibile, tragico e di urgente attualità nella cronaca quotidiana del nostro Paese, dove la forza drammatica degli eventi ha reso quasi inevitabile Un fenomeno aberrante contro il quale, insieme con la collega Mussolini, prima firmataria, e tante senatrici e senatori del Gruppo, abbiamo presentato un disegno di legge dal titolo chiaro ed inequivocabile: «Introduzione del reato di femminicidio». Questo è il salto culturale. Non norme astratte sulla violenza di genere, non norme astratte sulla violenza di un sesso contro l'altro, ma indirizzi mirati e più che mai necessari contro un fenomeno inquietante, odioso, terribile che va contrastato con norme chiare, specifiche e decise: non norme tese a contrastare una teorica violenza di un sesso contro l'altro, ma la violenza alle donne. Questo è il grande valore della Convenzione di Istanbul, questo è il grande valore di questa ratifica, che speriamo contribuisca ad una sollecita entrata in vigore. motivo di orgoglio per il nostro Paese il grado di prontezza e il livello di consenso con cui il Parlamento sta procedendo a segnare, auspicabilmente, una strada anche

prevenzione, protezione, perseguimento dei colpevoli e partecipazione. Mi compiaccio molto (l'ho già detto in apertura) dell'approccio chiaro e responsabile che la Convenzione adotta nei confronti del perseguimento della violenza contro le donne, la terza fare almeno un accenno alle prime due "p" non meno importanti, la protezione e la prevenzione, perché perseguire i colpevoli è fondamentale, ma da solo non può bastare. Così la Convenzione, tra le molte misure, stabilisce che si debbano finanziare con risorse pubbliche sia le organizzazioni non governative per la protezione alle donne sia il risarcimento alle donne che abbiano subìto violenza. È un impegno che non deve restare una buona intenzione. anche per la cronaca che spesso non dà il giusto rilievo a questa vera emergenza sociale. Basti ricordare l'ultimo episodio della sedicenne di Corigliano Calabro, riguardo al quale sono stati sottolineati gli aspetti Non deve restare una buona intenzione anche per la giustizia, perché una sentenza resa dopo troppi anni, anche se giusta, è essa stessa una forma di violenza. Le dichiarazioni del Ministro fanno ben sperare. Ma, in Parlamento voglio dar voce al dubbio che di recente ha espresso la consigliera nazionale di parità Alessandra Servidori: non è che creiamo delle aspettative di agire veramente sulla violenza e poi non ne abbiamo concretamente la possibilità? Su questo serve un impegno continuo, univoco e responsabile. Preferirei che noi tutti fossimo tacciati di *jusqu'au-boutisme,* (fino al limite delle nostre possibilità) termine che comprende una sorta di accanimento nel perseguire un obiettivo. Serve un salto di qualità delle istituzioni e di quella che viene definita la società civile. Uno sforzo che possiamo e dobbiamo fare tutti insieme perché diventi un sentire comune il messaggio che la violenza contro le donne è una inaccettabile violazione dei diritti umani. Si aggiungono ora nuove prove: le nuove sfide cui la Convenzione ci mette di fronte. Come potrebbe essere costruito il nuovo sistema di protezione delle vittime cui la Convenzione da particolare rilievo? Come saranno finalizzate le altrettanto rilevanti misure volte a colpire i matrimoni forzati, sempre più numerosi in tutta Europa, e non solo in Italia, che considero epifenomeni di un inaccettabile analfabetismo culturale di ritorno? In tal senso, mi sembra di grande interesse - non solo da un punto di vista tecnico - l'invito che la Convenzione rivolge agli Stati affinché nei procedimenti penali intentati a seguito di atti di violenza le motivazioni fondate sulla cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto onore non possano mai essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Ricordiamo con raccapriccio l'omicidio di Hina e le sue motivazioni. Di grande interesse, dicevo, questo aspetto, ancorché non adeguatamente valorizzato che ci dovrà spingere ad effettuare approfondimenti e dibattiti, anche se non vorremmo mai rinverdire antiche controversie su disposizioni che abbiamo faticosamente cancellato dai nostri codici (mi riferisco al cosiddetto delitti d'onore). Un aspetto, dicevo, delicato che dovremo trattare, perciò, con consapevolezza e senso di responsabilità, affinché quei valori di cui parlavo prima (cultura, usi, costumi e religioni) non scadano a principi interpretabili nel diritto e nelle coscienze, per non scivolare in un relativismo culturale e giuridico, quel relativismo culturale che vede, purtroppo, ancora presenti le mutilazioni genitali. Un invito a profondi cambiamenti di atteggiamenti e stereotipi culturali che tollerano, se non addirittura giustificano, tali forme di violenza. Dobbiamo lavorare, quindi, intensamente e senza risparmi affinché le donne, soprattutto quelle delle nuove generazioni, cancellino dal loro immaginario il sentimento della vergogna che impedisce loro di parlare, di raccontare la violenza subita, quella perpetrata da uomini che continuano a considerarla una manifestazione normale, il corollario di un tragico impulso di proprietà per un oggetto a loro estraneo ma, addirittura, molto vicino. Sappiamo che dare concreto seguito a questo impegno internazionale forse non sarà facile, ma è chiaro che la ratifica di oggi non è il termine di un impegno e non è il termine di un cammino, ma l'inizio. Con questo auspicio dichiaro il voto favorevole

signora Ministro, signora Vice Ministro, vorrei cominciare con un episodio. Ieri sera a San Giovanni al Natisone una donna è stata uccisa a coltellate dal marito davanti ai figli di otto e cinque anni. Lo dico perché credo che l'avvertimento lanciato dalla relatrice, senatrice Fattorini, di dover sfuggire ad una facile retorica di genere,

nel corso dei loro interventi - ed io condivido l'affermazione - che la violenza sulle donne e il femminicidio hanno natura strutturale perché ancora strutturale è l'elemento discriminatorio su cui si fondano; è la traccia e l'idea su cui si articola la Convenzione di Istanbul. Per essere più brutale, le donne si picchiano, si stuprano, si maltrattano, si offendono, si umiliano, si mortificano in quanto donne, perché si ritiene di operare secondo un naturale dominio su cui quei corpi, sulla base di una relazione gerarchica, che ammette solo sottomissione e non libertà; perché quelle donne quelle donne o quella donna sono proprietà, soggetto che si possiede; perché l'autonomia di quella donna è subordinata ad un potere naturale superiore; perché l'autonomia è in sé insubordinazione e oltraggio; perché le donne devono, esistono per accontentare gli uomini (sessualmente, ma non solo); perché se un uomo ama una donna ha diritto di averla alle sue proprie condizioni e di piegarla con la violenza a quelle condizioni; perché se una donna è legata ad un uomo (marito, amante, fidanzato) la disponibilità di quella relazione è solo nelle mani di quell'uomo e la libertà delle donne di troncare la relazione, affermando una libertà interiore e il diritto ad una relazione sentimentale soddisfacente, è arbitrio ed oltraggio. Perché il corpo delle donne, come ricordava la collega Bonfrisco, è continuamente proposto come luogo di scorreria degli sguardi e del desidero maschile, anche dai *media*, anche dai *media* colti di questo Paese, come se si trattasse di un'attrazione pubblica in un luna park; perché le donne devono tacere per interdetto tradizionale; perché picchiare una donna corregge quella donna ed è per il suo bene. Potrei continuare all'infinito. Perché, per queste ragioni, quella violenza non è legale, ma è in qualche modo legittima, cioè assistita da un consenso culturale; potrei dire in grande misura da un consenso sociale. Tutto questo non è che accade altrove. Accade ovviamente anche altrove nel mondo, ma accade qui in questo Paese ogni sacrosanto giorno: in questo Paese della cui civiltà giuridica e democratica siamo fieri; fieri; in questo Paese che ha questa Costituzione, questa storia, questo Parlamento. Succede qua anche più gravemente che altrove. Succede tra i nostri amici, tra i nostri conoscenti, tra i nostri parenti, tra i nostri colleghi. Succede qui, non altrove. Le colleghe hanno citato il numero degli assassini di donne in questo Paese. Ricordo molto brevemente: nel 2011 sono state uccise 127 donne e, per 7 donne su 10, c'erano stati precedenti episodi di violenza

7 milioni di donne - dico 7 milioni di donne - tra i 16 e i 70 anni, italiane naturalmente, sono state vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita: 7 milioni di donne! Dall'inizio degli anni '90 diminuisce il numero degli omicidi di uomini su uomini: aumenta esponenzialmente il numero degli omicidi di uomini su donne.

accordo trasversale tra donne. Citiamo con orgoglio, dunque, la nostra legislazione sulla violenza sessuale; sulla tratta degli esseri umani, e delle donne in particolare; sull'allontanamento del maltrattatore dal domicilio domestico, sullo *stalking*. Certo, siamo fieri di questa nostra attrezzatura normativa, ma evidentemente, se ancora ieri sera una donna è stata accoltellata a morte davanti ai suoi figli dal marito, non abbiamo fatto abbastanza; non abbiamo fatto ciò che andava fatto. *(Applausi dai

di straordinaria arcaicità: pensate alla riduzione in schiavitù, a fini sessuali, delle donne (abbiamo dovuto reintrodurre, modernizzandolo, il reato di riduzione in schiavitù, perché sembrava appartenere ad un passato così remoto da non riuscire a rintracciarlo nella nostra cultura giuridica e di legislatore). Ma ha, insieme, un dato di straordinaria modernità, perché l'uccisione di una donna oggi - che rimanda a riti arcaici e a culture primitive - ha in sé l'aspetto della straordinaria modernità della ragione per la quale si uccidono con tanta frequenza le donne, e le donne italiane: perché le donne italiane, sulla propria libertà, autonomia ed autodeterminazione hanno costruito in questi decenni uno dei fenomeni più vivi, importanti e vitali della società italiana. dall'incontro tra il primitivismo del possesso e dell'arretratezza culturale e la modernità dell'affermazione del sé delle donne che nasce la gravità, la diffusione e la crudezza

sbaglieremmo e gravemente, se affrontassimo la questione soltanto sotto il profilo penalistico, che è certamente importante, come diceva la collega Alberti Casellati: al riguardo c'è una proposta di legge

però anche un'altra questione essenziale, che è una questione politica di primo rilievo. I diritti delle donne sono diritti umani, e su questo ormai non penso ci possa essere più dubbio. Ne consegue che la loro violazione è violazione di diritti fondamentali, e la loro violazione conduce ad una responsabilità del nostro Paese di fronte alle istituzioni internazionali. L'Austria è stata appena condannata per non essere stata in grado di prevenire l'omicidio di una donna da parte di suo marito, sentenze della Corte internazionale. Questo significa che non basta un quadro normativo adeguato. Occorre, e occorre per davvero, che l'Italia presti vera attenzione all'applicazione di ogni norma e di ogni obbligo internazionale che riguardi la violenza sulle donne, ma occorre che questo venga a dimostrazione della qualità complessiva della presenza dell'Italia sullo scenario internazionale. Siamo molto attenti alle *performance* dell'Italia circa gli obblighi economici e finanziari che contrae nelle istituzioni sovranazionali, ma siamo troppo troppo poco attenti alle *performance* del nostro Paese quando si tratta di prestare ossequio agli obblighi che abbiamo assunto nella celebrazione e nell'affermazione dei diritti di libertà e dei diritti umani. Questo

ci vuole organizzazione, ci vogliono politiche, ci vuole verifica delle politiche. Che non accada mai più che l'Italia non risponda al questionario 2013 sull'implementazione delle politiche che riguardano la violenza sulle donne, questionario rivolto all'Italia nel corso dell'indagine da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. *(Applausi dai Gruppi* *PD, PdL e Misto-SEL)*. Un Paese si valuta non soltanto se rispetta i parametri economici e finanziari, ma se riesce ad essere il luogo nel quale gli impegni solenni, cui anche i Parlamenti dedicano tanta attenzione, attenzione, vengono verificati con la stessa accuratezza, con la stessa forza e, lasciatemelo dire, con lo stesso orgoglio, perché affermano la qualità democratica del nostro sistema, l'eccellenza dell'Italia nel panorama internazionale.

il Senato, con il voto finale del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul, sta per approvare un atto fondamentale per le donne. Un atto che, se ne saremo capaci, potrà davvero segnare un profondo cambiamento culturale e sociale nella vita della nostra società. Per questo, d'accordo con la ministra Idem e la vice ministra Dassù, propongo all'Assemblea

parlamentare, con un minuto di raccoglimento tutte le donne, le ragazze e le bambine che nella vita e nella morte hanno subìto violenza fisica o psicologica.

Mi scusi, senatore, può intervenire o per un richiamo al Regolamento o sull'ordine dei lavori.

se c'è un'incertezza sull'esito della votazione stessa. Ma nel caso specifico, poiché si trattava di una approvazione praticamente unanime, non vi era alcuna incertezza sull'esito e quindi la richiesta di controprova è

La controprova viene richiesta subito dopo la votazione. Lei non ha dato l'esito della votazione e non ha chiesto gli astenuti. Noi non abbiamo potuto votare, e vorrei che rimanga

Presidente, credo che il problema sia superato, dal momento che il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha modificato le sue richieste. Tuttavia, vorrei dire una cosa, signora Presidente, senza nulla togliere al suo intervento. La richiesta di controprova si connotava per una sua tardività, perché la controprova, come ella ben sa e come è prescritto dal Regolamento, richiede l'identità del corpo votante, tanto è vero che si procede alla chiusura delle porte. richiedere la controprova a distanza di diversi minuti, quando non vi è la certezza dell'identità del corpo votante, mi sembra essere una richiesta tardiva. Per il resto, se me lo consente, onde evitare per il futuro ulteriori incidenti ulteriori incidenti che probabilmente si rapportano a una non corretta lettura del Regolamento, vorrei ricordare a me stesso - come usavo dire nelle aule di giustizia - che, secondo il Regolamento,

Ciò equivale a dire, sotto il profilo del Regolamento, che non sono consentite richieste cumulative per tutte le votazioni, né la richiesta del voto elettronico può essere sostanziata esclusivamente da una piccola alzata di mano. La ringrazio. Questa è una rilevante e significativa differenza, come il senatore sa, rispetto al Regolamento della Camera, che rende forse

una collega di un altro Gruppo, la collega Bisinella, ha ricordato di aver lei stessa prodotto analoga richiesta. Se questa non è evidenza cartesiana, ci si deve spiegare che cosa sia. Noi riteniamo profondamente oltraggioso il comportamento di chi, facendo finta di non vedere, non dà alle minoranze e alle opposizioni la possibilità di esercitare il proprio diritto di farsi valere.

o dal Presidente, quando ritiene che, sulla base del risultato, ci possano essere dubbi sul novero dei voti, oppure su richiesta di un senatore

licenziato dalla Presidenza. Poiché abbiamo continuato ulteriormente a votare, mi pare che questa discussione debba essere definitivamente accantonata, per non perdere ulteriore tempo in quest'Aula.

osservazione o una scarsa evidenza delle richieste, perché non vi era alcun motivo per rifiutare la richiesta di voto elettronico.

quando questo sia stato richiesto; penso che, ferma restando l'esigenza di speditezza dei nostri lavori, questo atteggiamento sarà confermato nel prosieguo

rilevazione delle richieste non si ripeta in futuro. Mi auguro, quindi, che questo basti ai colleghi per essere rassicurati sul fatto che non si vogliono comprimere le prerogative dei singoli parlamentari né, tantomeno, dei Gruppi.

Presidente, non so quale sia il metodo per potersi iscrivere per intervenire: se devo togliermi la giacca, lo faccio volentieri. È evidente, che vi è una certa distrazione della Presidenza nel cogliere la segnalazione degli interventi dei colleghi. Io stesso da circa un quarto d'ora cerco di farle capire che vorrei dire la mia, per quanto riguarda il mio Gruppo, sull'argomento. Detto questo, invitando quindi ad una maggiore attenzione, richiederei ai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle di non utilizzare la richiesta del voto elettronico come impedimento alla celerità dei

abbastanza incredibile. Abbiamo fatto la prima votazione nominale sul recepimento della Convenzione di Istanbul: il ministro Idem

la ministra Idem non è intervenuta per non riaprire la discussione, anche per deferenza all'Assemblea, ma ha chiesto che fosse registrato il suo voto, quindi risulterà votante.

finalizzato a sviluppare politiche che aiutino a migliorare la qualità delle risorse di acqua dolce e ad individuare situazioni di crisi idrica. Questo programma mira a coordinare le azioni delle Agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di tale gestione. Il disegno di legge al nostro esame ratifica il Protocollo d'intesa relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, del *Programme Office on Global Water Assessment* da parte dell'UNESCO. Le ragioni per le quali a questo Protocollo si è pervenuti soltanto nel 2010 sono imputabili probabilmente a difficoltà con l'istituzione regionale, nel senso che che l'ufficio di Perugia ha avuto forse vicende travagliate negli stessi rapporti tra la Farnesina e la Regione Umbria. Fatto sta che il Protocollo, seppur firmato nel 2007, non è poi stato ratificato nel nostro Paese per le difficoltà di carattere economico-finanziario - suppongo - nel rapporto fra il Governo nazionale e la Regione umbra. Le ragioni per le quali gli uffici del Programma hanno potuto rimanere a Perugia hanno consentito un'ultima proroga soltanto fino fino al 31 dicembre 2012. Nel frattempo il nuovo negoziato fra l'Italia e l'UNESCO, che ha modificato i contenuti economici dell'accordo del 2007, ha portato al Protocollo d'intesa della cui ratifica abbiamo discusso in Commissione;

Il Protocollo si occupa in primo luogo del funzionamento del Segretariato, dello *status* di questo Segretariato e della sua amministrazione. Viene poi definito il contributo che il nostro Paese si impegna ad erogare all'UNESCO, che viene ridotto di circa un terzo (anzi qualcosa di più) rispetto al passato. del Protocollo vengono definiti gli obiettivi del Segretariato di Perugia, tra cui si segnala come particolarmente rilevante il rapporto sullo stato delle risorse idriche mondiali e il supporto agli Stati membri per la valutazione dell'efficacia dei programmi nazionali di politica idrica. Ci sono poi norme sulle attività congiunte

Oltre agli articoli che stabiliscono ratifica ed ordine di esecuzione del Protocollo, il disegno di legge reca, all'articolo 3, la copertura degli oneri derivanti, pari a circa 2.300.000 euro annui.

e ha una valenza scientifica rilevante. Vorrei sottolineare in particolare che la questione della gestione delle acque sul piano nazionale ed internazionale

proporvi un tema di riflessione più generale concernente il modo in cui gestiamo gli organismi internazionali. In questo caso viene riconosciuto che il Paese ospitante e finanziante (almeno in parte) un'attività internazionale ha anche il dovere e il diritto

Presidente, onorevoli colleghi, poche parole per anticipare un voto pienamente favorevole. Ringrazio il relatore, senatore Compagna,

tecnico-scientifiche, politiche e socio-culturali. Ed è abbastanza sconcertante - lasciatemi dire - che questo Programma internazionale, che gestisce e valuta le risorse idriche a livello mondiale e che è da cinque anni in Italia, non sia stato assolutamente considerato e messo in attenzione della stampa nazionale. Brevemente, vorrei illustrare i contenuti dell'accordo per gli aspetti più significativi. Un primo aspetto è la possibilità di incidere attraverso questa struttura negli indirizzi di politica, non solo per il tema delle risorse idriche, ma anche per quello dello sviluppo sostenibile, dando quindi al Paese, in termini di politica estera e di politica estera culturale, uno strumento potente in più. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare e che ha puntualmente richiamato la vice ministro

che non casualmente inserisce il tema delle potenziali attività congiunte. Io sono stata rettore all'Università per stranieri di Perugia nel 2007 quando è stato siglato il *trust fund*, che è l'inizio del percorso. Vi garantisco che il percorso è stato travagliato non solo per ragioni economico-finanziarie, ma anche perché con l'UNESCO si è dovuto arrivare a questa importante novità. una sede ospitante, ma siamo una sede che vorrà interagire sul piano scientifico, politico ed istituzionale. Quindi, questo è un successo della comunità accademica, della Regione umbra e del Governo italiano: cerchiamo di viverlo con tale spirito anche per il futuro.

la votazione nominale mediante procedimento elettronico perché c'è una tendenza, che va contrastata, ad usare le ratifiche come riempitivo del programma d'Aula e a relegarle in momenti di scarsa attenzione da parte di tutti noi.

esame è un Trattato internazionale importante, perché riguarda la decisione di collocare nel nostro Paese la sede di un Programma la sede di un Programma internazionale dell'UNESCO in ordine alla valutazione sulle acque, che rientra in un programma rilevante come quello che consente l'accesso a tutte le persone, a tutte le donne e gli uomini del pianeta, a un bene primario e fondamentale come l'acqua, e consente un utilizzo dell'acqua sostenibile dal punto di vista ambientale. Tutti comprendiamo quanto tale questione sia fondamentale per il futuro dell'umanità e quanto sia estremamente importante che l'Italia si sia conquistata il privilegio - che poi naturalmente è anche un onere finanziario - di ospitare in casa sua,

due Gruppi sono assenti. Questo è il vero oltraggio al Senato e al popolo sovrano, non l'aggettivo che hanno rivolto a lei per non avere visto la loro richiesta.

Oggi è il compleanno di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace, che compie 68 anni. Sono molto contenta che quest'Assemblea voglia farle giungere i nostri auguri, il nostro affetto, il nostro ringraziamento ed incoraggiamento per l'impegno che per molti anni ha voluto mettere in campo per portare il suo popolo alla libertà e per l'impegno che dispiega ancora per accompagnarlo in questo percorso verso la democrazia. Dalle elezioni del 2011, che sono state solo le terze in mezzo secolo di storia della Birmania, questo Paese è cambiato e c'è un nuovo inizio. Si è Si è insediato un Governo finalmente civile - almeno formalmente civile, anche se ne fanno ancora parte molti ex militari - che in due anni si è reso protagonista di aperture fino a quel momento impensabili: sono stati liberati prigionieri politici, è stata allentata la censura nei *media* e sono stati assunti accordi importanti con alcune minoranze etniche. Di questo cambiamento è protagonista anche l'Unione europea e al suo interno il nuovo presidente Thein Sein, è stato in Europa e anche in Italia nella scorsa primavera. Segnali di questo cambiamento sono anche le cancellazioni avvenute nello scorso mese di aprile della maggior parte delle sanzioni contro la Birmania, eccettuato l'embargo sulle armi, che ancora permane,

e c'è un problema fondamentale da superare nell'impianto costituzionale del Paese che impedisce ancora la piena e libera partecipazione alle elezioni presidenziali. Aung San Suu Kyi è in Parlamento, ma non può candidarsi alle prossime elezioni presidenziali perché una norma della Costituzione impedisce ai cittadini birmani che abbiano parenti stranieri di candidarsi alle elezioni presidenziali. Questa è evidentemente una norma *ad personam* che speriamo sia superata. La ricostituita associazione «Amici della Birmania», che già dal 2007 ha accompagnato all'interno del Parlamento italiano il percorso di Aung, vuole di

che riguarda la situazione di crisi dell'azienda Berco nel ferrarese. Lo chiedo oggi perché sono venuta a conoscenza del fatto che il Ministro interrogato risponderà ad un'analoga interrogazione domani alla Camera; interrogazione che è stata presentata più di un mese dopo rispetto a quella che abbiamo presentato noi qui al Senato. Sarebbe quindi importante che, come il Ministero domani risponderà alla Camera, voglia fare lo stesso nei confronti di quest'Aula.